L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il decreto-legge, della cui conversione oggi ci occupiamo, ritorna al Senato dopo che questo ramo del Parlamento lo aveva approvato nel suo contenuto originario, cioè l'accorpamento delle elezioni amministrative nella provincia dell'Aquila al turno ordinario di elezioni amministrative che si terrà nel 2010. Già in Senato si era posto un problema di più ampio respiro, cioè trovare una formula, una normativa (naturalmente condivisa nel modo più ampio possibile) che consentisse di abbinare e accorpare le elezioni amministrative

la finestra entro la quale tenere le elezioni amministrative, anticipandola dal 15 aprile al 15 marzo. Questo consentirà al Ministro dell'interno di fissare la data per le consultazioni amministrative in concomitanza con la data delle elezioni regionali. Faccio presente che, comunque, per le elezioni regionali rimane un problema di perché il meccanismo previsto per le elezioni regionali è tale da determinare ogni quinquennio un'anticipazione del turno elettorale. Tra un paio di quinquenni, se su questo

un ampliamento della finestra per le elezioni amministrative e prevede inoltre, al secondo comma dell'articolo 1-*bis*, due aggiustamenti per consentire, in base ai meccanismi di convocazione dei comizi (e, quindi, anche di svolgimento delle pratiche amministrative connesse al turno elettorale amministrativo), di potersi potersi attuare con i tempi necessari che la legislazione ordinaria prevede. Si anticipa quindi al 24 gennaio il termine - che ordinariamente era del 24 febbraio

in maniera approfondita, della situazione delicata e complessa che si è creata nella città dell'Aquila e nei Comuni del cratere sismico dopo il dramma del terremoto. Non vorrei quindi apparire come ripetitivo o affetto dalla mania di considerare la questione dell'Abruzzo pregiudizialmente prioritaria, ma così è. Noi dell'Italia dei Valori confermiamo quanto già dichiarato in occasione della prima lettura della conversione del decreto-legge n. 131, ossia la nostra condivisione piena e completa

autunnale, con condizioni climatiche totalmente avverse, era fantasia (per non usare altri termini che potrebbero esprimere un giudizio implicito

Gli uffici regionali sono entrati in tilt e si trovano in una situazione di crisi, perché vi sono 3 milioni di metri cubi di macerie, pari a 4,5 milioni di tonnellate complessive:

altrettanto drammatiche. È bene, allora, che l'Aula di questa importante istituzione sappia a chi ci stiamo rivolgendo quando

ci stiamo rivolgendo a 7.000 persone che sono ancora in tenda; a 20.000 cittadini aquilani e della Provincia dell'Aquila che sono stati dislocati sulla costa, ad un'ora e mezza di

a 16.500 lavoratori che sono in cassa integrazione, nonché ai titolari di 1.500 imprese piccole e medie, ancora ferme dal mese di aprile.

del clima di sfiducia che alberga nella popolazione dell'Aquila e della Provincia, Provincia, perché, nonostante fossero stati messi in atto dei provvedimenti logistici, come l'uso di trasporti dalla costa all'entroterra,

dimostra il clima di forte preoccupazione che vive la città dell'Aquila. Allora questo provvedimento, che - ripeto - per noi è un atto dovuto e un atto condivisibile da parte del Governo e da parte dei due rami del Parlamento, deve essere anche un'occasione per riflettere su queste cifre che ancora sono il segnale, il termometro di una situazione che non è assolutamente come quella che si vuole disegnare attraverso gli strumenti mediatici o attraverso inaugurazioni ad effetto.

si facesse carico di un problema che è stato sollevato da noi dell'opposizione, insieme ai colleghi del Partito Democratico, in più occasioni. A fine anno, ai cittadini che vivono questa situazione drammatica, se non vi saranno provvedimenti di proroga,

il pagamento delle bollette di gas, elettricità e acqua, il pagamento del bollo auto, la carta acquisti per la spesa alimentare. delle consultazioni elettorali, debba dare un segnale in questo senso per aiutare a recuperare la fiducia dei cittadini della Provincia dell'Aquila. Ritengo che questo sia un atto dovuto e da parte nostra staremo attenti perché si possano creare quei percorsi per arrivare ad una soluzione positiva.

che finalmente ci troviamo un decreto-legge con veri requisiti di necessità ed urgenza che possiamo votare. Le altre due sottolineature sono le seguenti. Come ha accennato prima il senatore Pastore, al di là di come risolviamo *una tantum* il problema dell'*election day*, abbiamo un problema di slittamento progressivo a ritroso delle elezioni regionali, dovuto all'applicazione dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, che prevede che le elezioni dei consigli regionali si debbano svolgere nelle quattro settimane che precedono la regolare scadenza del quinquennio. Cosa è accaduto? Pur essendo transitata la competenza alle Regioni, di fatto si continua ad agire dentro questa norma. Quindi - do solo i dati - abbiamo votato nel 1970, nel 1975 e nel 1980 nel mese di giugno;

nel 2005 al 3-4 aprile ed ora siamo arrivati all'ultima domenica di marzo. Io penso quindi che il Governo e le Regioni dovrebbero stabilire insieme un tavolo istituzionale per evitare che di questo passo tra 5, 10, 15 anni ci si trovi ad aprire le urne a Natale, perché questa è la deriva naturale del meccanismo che abbiamo scatenato. Infine, vorrei sottolineare che

il tetto di due mandati anche per i Presidenti di Regione: si tratta di interpretare la norma. Tra l'altro, nei siti Internet di diversi giuristi si confrontano varie teorie sul se e quando la legge entrerà in vigore, il che incide, evidentemente, sull'elettorato passivo dei candidati uscenti. Ora, ad avviso prevalente, essa sarà operante dal 2015 perché, non potendo essere retroattiva, i mandati si conterebbero dal 2005. Tuttavia, per avere certezza del diritto ed evitare impugnative dei risultati elettorali, sarebbe bene che il Governo desse anche la sua autorevole opinione.

convertito qui al Senato, accogliendo, come ha ben illustrato il relatore, l'ulteriore modifica apportata dalla Camera.

al quale si sta cercando di portare riparo più velocemente possibile. Si è sbagliata l'impostazione iniziale, che è da ascrivere unicamente alla responsabilità del Comune dell'Aquila. Per quanto riguarda i disagi degli aquilani, vorrei ricordare a tutti

appartamenti con tutti i comfort necessari. Credo che criticare la gestione dell'emergenza all'Aquila sia veramente pazzesco ed inaccettabile.

un giornalista e un'attivista di un'organizzazione ambientalista) vengano espulsi da un Paese e privati dei loro diritti soltanto perché erano andati a verificare la situazione delle foreste.

tramite, signora Presidente,

che sono in affitto da lungo tempo. La gestione dei soldi degli agenti di commercio, investiti in prodotti derivati e in titoli Lehman,